prevedere, già nella delega, che gli interventi in materia di fiscalità di sviluppo, che sono stati introdotti dalla lettera *hh)* al comma 2 dell'articolo 2, comprendano due strumenti che sono stati già utilizzati e che, se precisati, al di là degli altri interventi in materia di fiscalità di sviluppo che possono essere adottati per le aree più disagiate del Paese,

considerato che in relazione ai principi specifici indicati all'articolo 2 relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali delle autonomie locali si fa riferimento "alla autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva.", ribadisce che tale riferimento non intende interferire nelle materie proprie della contrattazione, anche per evitare che il "costo del lavoro" possa divenire oggetto di competizione impropria tra le diverse Autonomie al fine della determinazione dei costi *standard*, conferma la volontà di valorizzare la contrattazione di secondo livello nell'ambito delle Autonomie, per incrementare quantità e qualità dei servizi intervenendo su temi quali la produttività, l'organizzazione del lavoro, le professionalità.

pregare non solo il relatore ed il Governo, ma anche i colleghi di prestare un momento di attenzione. Uno degli elementi critici - che abbiamo sottolineato con forza - del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri

troppo ampi. Non vi è alcun dubbio che il testo che stiamo esaminando oggi abbia significativamente ristretto l'ampiezza di questo eccesso di discrezionalità, che secondo noi presentava addirittura profili di illegittimità costituzionale: oggi, il disegno di legge - che pure non ci soddisfa pienamente, anche sotto il profilo dell'ampiezza della delega - sicuramente è più ristretto. Un altro dei punti qualificanti che avevamo sottolineato, però, era il fatto che esso - rispetto ad un meccanismo come questo, che comunque prevede che una parte fondamentale dell'esercizio della funzione legislativa sia svolta dal Governo

l'ambito di tempo era molto limitato e l'efficacia del controllo parlamentare obiettivamente troppo ridotta. è la ragione per la quale i senatori del Gruppo del Partito Democratico - ma, devo dire, sostenuti anche da altri senatori, tanto dell'opposizione quanto della maggioranza - hanno formulato una precisa richiesta, tendente

con il compito specifico di esaminare con pienezza di funzione il testo dei decreti legislativi. Diamo atto al Governo - nella fattispecie, al ministro Calderoli, ma anche al relatore Azzollini - di aver accolto questo principio: credo che oggi si possa dire che il nuovo articolo 3 è sicuramente uno dei passi in avanti più importanti che hanno hanno modificato l'impianto complessivo del testo di legge che stiamo esaminando. Ovviamente, non possiamo che confermare la soddisfazione per questo punto significativamente riconosciuto. Abbiamo però presentato egualmente, signor Presidente, un emendamento, il 3.1, che riscrive il testo approvato dalla Commissione e vorrei brevemente illustrare ai colleghi quali sono le due più significative differenze. una di queste differenze riguarda la composizione della Commissione. Il testo approvato dalla Commissione prevede che la Commissione sia composta esclusivamente da parlamentari; il lavoro, quindi, viene svolto secondo la consuetudine dei lavori delle Commissioni parlamentari e viene costituito, al fianco della bicamerale, un organismo del tutto separato cui partecipano rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e delle Province.

esclusiva dei parlamentari a esprimere il voto, affermi la partecipazione in maniera utile anche per la Commissione parlamentare dei rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni

L'altro punto, che forse è ancora più importante per noi e che differenzia il nostro emendamento da quello presentato e approvato dalle Commissioni l'efficacia del parere che le Commissioni esprimeranno. Mentre sotto questo profilo il testo delle Commissioni riunite non si differenzia dalla tradizione dei pareri espressi dalla Commissione - in fondo la novità sta nel fatto che si tratta di una Commissione bicamerale che si occupa esclusivamente di questo punto - nel testo che noi proponiamo viene prevista la possibilità, qualora il Governo non

non una norma costituzionale in senso tecnico, ma la previsione del federalismo fiscale ha i crismi dell'attuazione di una previsione costituzionale.

una Commissione bicamerale che abbia intanto una durata stabile, perché il controllo parlamentare sul federalismo e sull'attuazione del federalismo fiscale non inizia e finisce con i decreti attuativi. È evidente che questa materia stravolge in maniera permanente i rapporti finanziari e istituzionali tra Stato, Regioni ed autonomie locali. Vi è, pertanto, la necessità che vi sia una Commissione *ad hoc* che verifichi, monitori controlli se le cose che ci sono scritte o che verranno scritte nei decreti attuativi avranno un loro ancoraggio ai principi che questa delega generalissima sta dando.

alle funzioni, alle competenze e al ruolo di questa bicamerale e, quindi, dovrebbero essere assorbite e trasferite in questa bicamerale permanente che si occupa di questo tema. L'idea che si possa istituire una Commissione a tempo, con poteri limitati, in realtà cela un altro intento - mi dispiace non essere d'accordo con il collega Bianco

dei decreti attuativi, non avrà alcun controllo diretto sulla gestione complessiva e sulle politiche che lo Stato, le Regioni e il sistema delle autonomie avranno in materia. A svolgere tale

questi, infatti, sono compiti propri dell'attività parlamentare. Torno a dire - sarò noioso, signor Presidente - che l'articolo 119 della Costituzione, sul fondo perequativo e sulle risorse che riguardano le aree sottoutilizzate del Paese, non può essere espropriato, norma costituzionale. È questa la sede in cui si compie la sintesi legislativa e politica delle istanze del Paese, soprattutto con riferimento al fondo perequativo e al fondo per la coesione sociale. questa competenza, introducendo una sorta di Conferenza Stato-Regioni e autonomie parallela è un modo per anticipare fuori dai confini della Carta costituzionale

Senatore Zanda, ogni riferimento a fatti attuali è puramente casuale!

apprezzato maggiormente la stesura letterale del nostro emendamento, ma non si può non riconoscere che il testo che viene messo in votazione

Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto. Il Gruppo dell'Italia dei Valori, nel corso della lunga discussione in Commissione, aveva presentato una proposta leggermente diversa da quella che poi è stata scelta.

Ritenevamo che questa fosse una soluzione efficace per aumentare l'efficienza della Commissione e realizzare minori sprechi. Prendiamo atto del fatto che è stata adottata un'altra soluzione. Preferivamo la nostra, ma il realismo vuole che ci si confronti con una proposta che è passata per convinzione della maggioranza. Voteremo pertanto a favore, ricordando che avevamo cercato un cammino analogo, ma a fianco

si dovrebbe tornare alla situazione originaria prevista dalla prima composizione. Vorrei porre alla sua attenzione, visto che lei ha fatto una glossa

dando la possibilità ai Presidenti dei Gruppi o ai capi di partito di modificare o alterare le loro rappresentanze rispetto ad un voto del Parlamento,

che sono nominative, non piacessero più, in una data successiva, a questo o a quel Presidente di Gruppo parlamentare o a questo o a quel segretario di partito, la volontà del Parlamento,

se questo non sia un altro dei tanti casi cui assistiamo in questi ultimi anni di una diminuzione del valore e della funzione, non voglio dire del prestigio, del Parlamento, come se questo non fosse un organo costituzionale e, invece, fosse più importante e certamente prevalente l'organo politico che è estraneo al Parlamento medesimo.

Presidente, lei, interrompendo il presidente Pera, ha parlato di caso di analoga attualità. Credo che a questo punto si dovrebbero sospendere i lavori e analizzare quale sia questa analoga attualità,

regola sovrana della nostra democrazia, vale a dire sono i Gruppi parlamentari che indicano i senatori che partecipano alle Commissioni e tali indicazioni devono essere perfettamente aderenti alla proporzione

dal punto di vista proprio dell'ordinato svolgimento dei lavori e degli equilibri politici che sono necessari e costituiscono la natura della nostra attività di parlamentari,

Credo che ciò non abbia nulla a che vedere con la prescrizione della Costituzione che dà a ciascuno di noi doverosamente - e personalmente ne sono uno strenuo difensore - l'assoluta libertà di mandato, che si estrinseca

di acquisizione, di accertamento, per cui c'è la necessità che la legittima esigenza della proporzionalità sia contemperata con l'altra esigenza costituzionalmente garantita, che è quella del divieto di mandato imperativo. questione sia quella della Giunta. La seconda ragione, che non è certamente nelle intenzioni del collega Zanda, ma può essere attribuita all'intenzione di qualcun altro, è che a noi non piacciono le vendette postume. vorrei che non dessimo per scontata, al di là della motivazione di merito su questo singolo caso, l'interpretazione costituzionale che ha proposto il presidente Pera, perché nella nostra Costituzione, come nelle Costituzioni coeve, c'è una tensione tra due princìpi: da una parte vi è l'articolo 67, il divieto di mandato imperativo che ci deriva dagli Stati liberali presuffragio universale, che noi abbiamo giustamente mantenuto; dall'altra, vi è la linea di princìpi che va dall'articolo 1, che afferma nettamente la sovranità popolare, all'articolo 49, per cui i cittadini, attraverso i partiti, determinano la politica nazionale. I suddetti due principi sono in tensione tra loro e noi dobbiamo, volta a volta, decidere se ci pare più opportuna un'interpretazione che parte dagli articoli 1 e 49, che richiede quindi una costante fotografia dell'Aula nelle Commissioni, per cui l'articolo 67 è solo recessivo e riguarda il diritto del parlamentare a non decadere dall'Aula; diversamente, se partiamo dall'articolo 67, riteniamo dominante detto articolo e recessivi gli articoli 1 e 49.

Non credo che si possa rinviare la questione alla riforma del Regolamento, perché il Regolamento riguarda solo le Commissioni monocamerali. Qui siamo in presenza dell'istituzione di una Commissione bicamerale *ad hoc*, quindi in questo caso dobbiamo decidere quale delle due linee meglio si adatta a tale Commissione bicamerale.

penso che quest'Aula debba essere grata al riferimento implicito al caso di attualità, fatto da lei con grande eleganza, e

A che cosa ci si riferisce? Alla proporzione di inizio legislatura? In tal caso, è chiaro che la norma è troppo *hard*, perché una democrazia parlamentare che presuppone il riferimento proporzionale fra i Gruppi al principio della legislatura è troppo rigida e fa troppa pressione sull'articolo 67. Se invece il riferimento dell'emendamento Zanda ha la caratteristica di

ha il limite formale che si rischia di non abbracciare le Commissioni bicamerali; ciò nonostante, le preoccupazioni che sono state espresse

un maggior rispetto formale dei principi propri del parlamentarismo e della libertà dei singoli parlamentari. Basterebbe eliminare dal testo dell'emendamento

Quindi, sostanzialmente, senatore Zanda, resta salvo il principio della sua proposta e

elimina l'inciso «su designazione dei gruppi parlamentari», ma lascia intatta l'ultima frase che recita: «la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari anche dopo la sua

sarebbe stata definita partitocratica; oggi invece si definisce *bipartisan*. La sostanza non è cambiata

o di un Segretario di partito politico prevalga sulla volontà istituzionale del Parlamento.

Questo è il principio che viene statuito dall'emendamento Zanda. Il senatore Zanda vuole questo per evitare la replica di quella che lei ha chiamato la giurisprudenza recentissima e che io definirei calda e caldissima. Vorrei far osservare, signor Presidente, che se si viola la Costituzione, la circostanza che essa venga violata in modo *bipartisan* non elimina il fatto che si consumi una violazione. Quello che stiamo facendo qui oggi è una violazione ha facoltà. FINOCCHIARO *(PD)*. Le confesso, Presidente, che nonostante l'autorevolezza degli interventi del presidente Pera, io non comprendo dove verrebbe violata la volontà istituzionale del Parlamento. Accade continuamente che ci siano voti in dissenso da parte di parlamentari che appartengono a ciascun Gruppo, e ce ne saranno su questo provvedimento. appartiene alla naturalità dell'esercizio della funzione parlamentare che nessun Gruppo parlamentare ha mai sconfessato, adeguando

da parte dei Presidenti di Camera e di Senato - peraltro in un organismo di garanzia in cui il rispetto della proporzionalità nella composizione assume un valore forse più alto di quanto non accada nelle Commissioni permanenti non vi è possibilità di dissociazione, ovviamente, che venga contemplata nei regolamenti come causa di espulsione. Ci potrebbero essere comportamenti che si pongono gravemente in dissenso rispetto ai singoli regolamenti e, in tal caso, i Gruppi parlamentari e i partiti di appartenenza decideranno, ipotesi peraltro del tutto eccezionale, mentre ipotesi assolutamente ordinaria, come abbiamo visto anche nella scorsa e nelle precedenti Legislature, è quella che un parlamentare, designato da un partito, cambi partito e Gruppo parlamentare. L'unico valore istituzionale da garantire, a questo punto, è che la proporzione nella rappresentanza dei Gruppi venga mantenuta inalterata dall'inizio alla fine del funzionamento dell'organo,

dei principi che devono governare il funzionamento delle Commissioni parlamentari: la libertà di esercizio della funzione parlamentare e, ovviamente, l'autonomia del Parlamento medesimo dai partiti.

Presidente, colleghi, ho ascoltato l'intervento della presidente Finocchiaro. Mi pare veramente un po' balzana l'idea di non passare per i Gruppi parlamentari. Se questa è una Commissione nuova stiamo inventando delle procedure diverse, facciamolo anche! Però non mi pare che sia questa la sede per innovare in maniera così radicale e di fatto stracciando tutta la scienza del precedente. Quindi, ritengo che l'emendamento

Innanzitutto, ringrazio il presidente Pera per aver risposto alla domanda che avevo posto a lei. Non si capisce però perché non si possa utilizzare l'articolo 21 del nostro Regolamento per la composizione di questa Commissione come avviene per tutte le altre Commissioni permanenti;

Poiché attraverso questo disegno di legge delega stiamo mettendo mano in maniera radicale e sostanziale a tutti i meccanismi di spesa pubblica, riteniamo sarebbe molto utile istituire una conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Abbiamo assistito in questa sede ad un "balletto" tra

Nel momento in cui si mette mano a tutto il sistema della spesa pubblica pensiamo che una conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sarebbe importantissima (in conclusione arriverò a dire che il Governo, nei fatti, dovrà farla).

esempio, a tutto il problema dei criteri attraverso i quali si andranno ad individuare gli standard dei servizi pubblici nel nostro Paese. È uno dei meccanismi fondamentali che sta alla base di questa legge.

li metta a punto, eserciti il controllo e renda disponibile un'interpretazione corretta dei dati per arrivare all'individuazione degli standard. Lo stesso si potrebbe dire per i livelli essenziali delle prestazioni nei Di fatto, il Governo sarà costretto non soltanto a convocare la Conferenza Stato-Regioni, ma a convocare Regioni, Comuni e Province ogni volta che dovrà fare questo tipo di lavoro, per allora non farlo attraverso la legge individuando una sede più autorevole, che metta in condizioni il Governo di porre in essere questo lavoro di armonizzazione della spesa pubblica e di interpretazione unitaria dei criteri per l'individuazione degli standard

che avremmo potuto utilizzare in altro modo e più proficuamente.

dell'utilizzo del fondo perequativo, ma anche di verifica periodica dell'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo. Proprio per questo riteniamo insufficiente che la Conferenza permanente metta a disposizione

tutte le informazioni che la Conferenza permanente possa raccogliere per rendere efficaci le sue funzioni pregnanti.

Presidente, questo emendamento sembra essere stato recepito, perché si ritrova inserito all'articolo 25,

Il tema è questo: il cittadino si troverà davanti a tributi comunali, provinciali o di città metropolitane, regionali, dello Stato; e il rischio che il mancato coordinamento di questi sistemi impositivi possa aumentare la pressione fiscale costituisce una preoccupazione seria.

di tutti i livelli di governo: questo è il fatto positivo. Inserire questa prescrizione nell'articolo 25, invece, costituisce un auspicio generico, che esclude sostanzialmente dall'individuazione della pressione fiscale massima i rappresentanti degli altri livelli di governo. In più, non è prevista una programmazione pluriennale dei livelli massimi di imposizione fiscale, un'assoluta necessità: oltre a prevedere il livello massimo d'imposizione fiscale, la Conferenza dovrebbe individuare la

forse si è distratto un attimo: lo capisco, dopo aver passato tanti giorni ad occuparsi di questi commi. Intervengo dunque io in dichiarazione di voto su questo emendamento, che considero particolarmente rilevante e che forse abbiamo avuto il torto di non illustrare in sede di illustrazione degli emendamenti. Signor Presidente, signor relatore, signor Ministro, noi proprio con l'articolo 17, cui il Ministro ha fatto adesso riferimento, abbiamo inserito in Commissione rispetto al testo del Governo

naturalmente al netto dell'oscurità della definizione, in buona sostanza consente sistematicamente di introdurre a fianco al concetto di fabbisogno standard relativo alla copertura dei costi standard dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi *ex* lettera *m)* del 117 della Costituzione il principio secondo cui ci sono anche fabbisogni ottimali di riferimento, in termini di quantità e qualità dei servizi, che via via in una logica pluriennale debbono essere precisati al fine del loro progressivo conseguimento vorrei dire al relatore e al Ministro - ai fini della verifica del loro mancato perseguimento (in una situazione nella quale evidentemente il patto di convergenza per alcune Regioni potrebbe non funzionare), in modo da definire le conseguenti iniziative volte ad affrontare il problema costituito dalla mancata convergenza. È un po' lo stesso meccanismo che si applica - signor Presidente, non è il caso che mi soffermi sul punto - in sede europea quando di fronte al patto di stabilità e crescita si manifestano comportamenti o andamenti divergenti nei singoli Paesi. Ora, noi cosa proponevamo di dire con l'emendamento 5.700? In coerenza con l'articolo 17 proponevamo che in sede di Conferenza, quella trattata nell'articolo 5, la verifica riguardasse anche gli obiettivi di servizio, in modo tale che la pluriennalità del patto di convergenza fosse sistematicamente verificata di anno in anno in sede di Conferenza. semplicemente di un emendamento la cui mancata approvazione introdurrebbe un equivoco riguardo alle competenze della Conferenza in rapporto all'introduzione dell'articolo 17.

che deve avere una sua dimensione e composizione su scala nazionale, intervenire con un eccesso di frammentazioni e di modulazioni possa in qualche modo rispondere, certo, all'esigenza di finanziare delle funzioni, ma correre il rischio di determinare effetti di natura regressiva e tali da inficiare la progressività ed unitarietà del tributo stesso. Da questo punto di vista, è vero ciò che ha detto il ministro Calderoli e cioè che già oggi esistono meccanismi per cui ci sono ampi margini di intervento sulle aliquote addizionali da parte del sistema delle Regioni, ma questa non è una buona motivazione. Noi, infatti, stiamo ridisegnando un sistema nel suo complesso e dovremmo cogliere tutte le opportunità per poter andare nella direzione di semplificare il sistema e di avere elementi di chiarezza e di leggibilità e non elementi che in qualche modo possano contribuire a rendere complicata l'interpretazione e l'applicazione delle norme e, soprattutto, poco trasparente per il cittadino l'allocazione delle responsabilità in ordine ai criteri

7.503 proponiamo una semplificazione di ordine lessicale. al posto dell'espressione: «propri derivati», preferiamo la formula «derivati», così da rendere evidente la distanza con i tributi propri, che sono invece quelli di iniziativa regionale. lettera *b)*, si affiancano, alle aliquote riservate alle Regioni, le addizionali, che rispondono alla medesima logica impositiva e di valorizzazione delle autonomie.

delegato un margine di discrezionalità troppo indefinito nella selezione dei tributi su cui ammettere un margine di autonomia regionale. Il Gruppo dell'Italia dei Valori apprezza l'accoglimento della sua proposta di salvaguardare l'osservanza del diritto comunitario. Segnalo di passaggio che comunque questa osservanza non può essere prevista solo per i tributi derivati, ma deve valere anche per quelli propri, ragione per cui abbiamo proposto anche un emendamento in tal senso all'articolo 2.

che in una legge di sistema come questa che è in discussione i criteri di territorialità dei tributi non possano essere previsti solo per i tributi derivati e le compartecipazioni, ma debbano necessariamente riguardare anche tutti i tributi regionali.

di sottolineare che sia per il punto n. 1 che per il punto n. 2 la Regione, attraverso un'apposita legge, ha facoltà di ampia modulazione e di manovra su questi tributi;

di deduzioni e così via che vanno ad incidere sulla determinazione della base imponibile. Questo per un'ottima ragione, che non è quella sulla quale si è soffermato anche stamattina il ministro Calderoli, ossia che ci sarebbe un'obiezione di principio al fatto di avere diversi sistemi IRPEF, perché, com'è stato ricordato, già con l'addizionale funziona così.

di tutti i tributi che questa legge dovrebbe proporsi di riordinare, assegnando con chiarezza, a funzioni diverse e istituzioni diverse, tributi diversi.

ce l'hanno solo sull'addizionale. Noi creiamo un contesto completamente diverso e in questo contesto l'IRPEF è un tributo nazionale, è un tributo dello Stato. Quindi, grande flessibilità e capacità di intervento sulla parte di scelta dell'aliquota da applicare nell'ambito della legge definita dallo Stato, ma nessuna modifica della base imponibile, perché questo renderebbe difficile poi la previsione centrale anche per il fondo perequativo.

tende a precisare, così come fatto in altri emendamenti, che ovviamente sono stati bocciati dalla maggioranza, il rispetto della struttura e dei principi di progressività di ciascun tributo. Anche quando sono di competenza regionale e/o locale, anche quando riguardano l'autonomia ampia che si dà ai Comuni, alle Province,

il criterio di riparto del gettito derivante dalla suddetta imposta non è dato dal valore aggiunto che quell'attività produttiva determina in quella specifica Regione, ma dal costo del lavoro. Da ciò deriva un'iniquità sotto il profilo del gettito fiscale che in questa sede sarebbe opportuno, almeno in via di principio, correggere, in modo da consentire

Io sospendo la seduta per dieci minuti.

Senato non approva.**

del sistema fiscale a proposito di una tassa di tipo erariale che noi consideriamo fondamentale, cioè l'IRPEF, che nei fatti prevede le aliquote, le addizionali

grossa parte dell'aliquota erariale, cioè dell'IRPEF, come unica tassazione statale sulla quale non agire con le manovre. la preoccupazione che si possano creare diversi sistemi di IRPEF regionali resta in noi ancora molto forte e, nonostante l'apprezzamento per il lavoro svolto, il nostro è un voto contrario politicamente, e vogliamo

è superato perché dal testo sono scomparsi i termini di assistenza, istruzione e sanità. Pur conservando il suo valore ideale, lo ritiro

il settore importante e strategico del trasporto pubblico locale ai livelli essenziali, garantiti al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, lettera

per cui il Governo garantiva per il trasporto pubblico locale soltanto un funzionamento adeguato nella proposta delle Commissioni, attraverso un'opera di mediazione, si è cercato di portare l'utilizzo del fondo perequativo del trasporto pubblico locale solo per garantire un livello di servizio minimo. L'emendamento ha il compito di riportare un po' di chiarezza tra queste due categorie, quella della totale copertura attraverso il fondo perequativo dei livelli essenziali, che comprendono sanità, assistenza e istruzione, e la e la terzietà del trasporto pubblico locale, di cui viene garantito tramite il fondo perequativo soltanto un livello minimo; perequativo soltanto un livello minimo; l'emendamento propone il riferimento e quindi il vincolo ai livelli essenziali di assistenza anche per il trasporto pubblico locale.

il Governo ad accogliere questo emendamento, e, laddove dovesse essere di difficile applicazione, cosa che non credo, eventualmente ad accettarlo come ordine del giorno, finalizzato a quello che sarà il confronto tra

l'emendamento 8.522 riafferma il principio proposto in seno all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, per ribadire in modo netto la necessità di limitare il ricorso alle compartecipazioni, viste quale strumento opaco

Dopo le parole: «diritto allo studio», considerando la carenza dell'edilizia scolastica e della formazione professionale, noi proponiamo

concetti. Bisogna prevedere sicuramente quanto egli richiede, ed è la nostra stessa preoccupazione, però occorre verificare di non andare ad aggravare ulteriormente una procedura che porta alla definizione dei che diversamente non consentirebbe quella adeguabilità che in certi momenti è necessaria e che attraverso procedure troppo complesse rischierebbe di rendere fuori tempo le variazioni.

chiediamo che il trasporto pubblico locale sia inserito fra i servizi essenziali ed i livelli essenziali delle prestazioni da indicare. La vera differenza tra l'attuale allocazione del tema del trasporto pubblico locale e quella che proponiamo con l'emendamento 8.534, che chiede l'inserimento all'interno del comma 2 dell'articolo 8, è appunto di evitare la differenziazione, oggi presente,

ma prevedendo, nel disegno di legge governativo come modificato, che le spese in conto capitale vedano la propria perequazione sul fabbisogno standard (e quindi al cento e quelle invece correnti sulla capacità fiscale. Ora, capite che inserire un servizio così importante come il trasporto pubblico locale fra i livelli essenziali delle prestazioni cambia radicalmente il livello di qualità del servizio offerto ai cittadini in tutto il Paese.

dall'emendamento 8.534 questo tipo di intervento farebbe sì che questa funzione diventi letteralmente importante per i servizi resi alle Regioni. Invito i colleghi senatori a ragionare bene, perché, una volta che non inserissimo il trasporto pubblico locale tra i livelli essenziali della prestazione, ci troveremmo in una giungla di servizi pubblici da distribuire.

Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto di astensione del Partito Democratico in quanto in questo articolo, che è assolutamente fondamentale perché riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali della Regione, ci sono delle mancanze. Ricordo, peraltro, che molti degli emendamenti che avevano presentato non sono stati raccolti; quello che però vorrei evidenziare è che invece sono stati fatti dei passi in avanti molto rilevanti rispetto alle

dalle Regioni e dalle autonomie locali. È stato, peraltro, accolto dal relatore e dal Governo un emendamento importante presentato dal senatore Barbolini, l'8.533, che apre comunque, sul tema dell'istruzione, la possibilità, attraverso intese fatte tra Stato e Regioni, di allargare il sistema degli interventi e delle competenze regionali su questa materia. È stato poi inserito il diritto allo studio, che mai era stato individuato come una funzione fondamentale dello Stato, finanziato attraverso i LEP. Questo determinerà una maggiore omogeneità e una maggiore opportunità per tutti i ragazzi nei diversi territori nazionali. Pensiamo che il diritto allo studio non attiene solo all'accesso all'istruzione, ma anche al successo scolastico e formativo e, quindi, è determinante. quello che, peraltro, ci aveva segnalato il sistema delle autonomie locali. Non viene individuata come competenza regionale, perché così non è nell'ordinamento attuale, e

un altro punto importante acquisito. Devo poi sottolineare, in sintesi, il nostro giudizio sull'ampia discussione che c'è stata sul trasporto pubblico locale. Il Partito Democratico ha sostenuto con grande determinazione e forza che il trasporto pubblico locale dovesse essere collocato tra le funzioni soggette ai LEP e, quindi, integralmente finanziate. Devo dire che la soluzione a cui siamo addivenuti costituisce un passo in avanti molto rilevante anche rispetto all'intesa assunta tra il Governo e le autonomie locali nella quale non era previsto il trasporto pubblico locale come sistema finanziato a LEP. Aver scelto qui di finanziare comunque a LEP gli investimenti per il trasporto pubblico locale e aver precisato, nelle competenze di Comuni e di Province, che quel trasporto pubblico locale costituisce una delle funzioni fondamentali finanziata a costo standard mi sembra rappresentare un elemento decisivo, sia per quanto riguarda la spesa per investimenti sia per quanto riguarda (la soluzione non è quella che noi avremmo voluto, ma è un importante passo in avanti) la spesa corrente. Rimane infatti, anche da conti che abbiamo provato a fare, una quota non molto rilevante di spesa regionale non finanziata a LEP. Per queste ragioni, ovvero per le carenze, da un lato, ma anche per i grandi miglioramenti, dall'altro, il nostro voto - come avevo preannunciato - è di astensione.

uno degli elementi di maggiore differenziazione tra la nostra posizione e quella del Governo e della maggioranza su un punto importantissimo che riguarda i meccanismi di alimentazione La discussione, come è noto, parte dal confronto polemico sul cosiddetto modello lombardo e, a seguito del confronto in Aula, è approdata l'affermazione del principio della verticalità del fondo perequativo, così come da noi richiesto. Senonché il Governo e la maggioranza si attestano su una posizione di alimentazione del fondo mediante la compartecipazione all'aliquota IVA. È questo uno dei punti di dissenso che con questo emendamento si intende superare. Infatti, è del tutto evidente che, attraverso questo meccanismo che tende a

il carattere orizzontale della perequazione, peraltro determinando un meccanismo che non garantisce la congruità del fondo di perequazione. Noi invece riteniamo che il fondo perequativo debba essere alimentato con la fiscalità generale, perché questo meccanismo è quello che garantisce l'adeguatezza del fondo stesso e il carattere effettivamente verticale della perequazione medesima. neanche il meccanismo di alimentazione del fondo basato sulla capacità fiscale, così come è congegnato nel testo approvato dalle Commissioni riunite, garantisce l'adeguatezza del fondo, soprattutto relativamente al finanziamento delle delle funzioni non essenziali e delle prestazioni non LEP, uno dei punti importanti che noi invece intendiamo affrontare nel modo in cui lo si affronta nel testo dell'emendamento 9.502, cioè garantendo che anche quelle prestazioni e funzioni possano godere di una quindi, il Governo e il relatore a porre attenzione su questo aspetto perché dall'approvazione di questo emendamento dipende anche una valutazione del provvedimento nel senso di una completezza e di una certezza dei meccanismi di un fondo, quello perequativo, che costituisce uno degli uno degli architravi di un edificio che altrimenti sarebbe destinato nel tempo a crollare.

delle Regioni è diverso dall'attribuzione del fondo perequativo che le Regioni danno ai Comuni. Mentre per i Comuni, giustamente, questo disegno di legge ha previsto che vengano considerate situazioni particolari, come le fasce altimetriche o l'invecchiamento della popolazione, per le Regioni si prende a base il costo standard. Stiamo facendo un errore enorme. federalismo, signor Ministro, e gliel'abbiamo dimostrato in tanti modi, anche perché per noi il federalismo è un nome, come ho spiegato ieri: in realtà, vogliamo lo Stato delle autonomie e il rispetto dei livelli dei livelli di potere locali. Ma come si fa, una volta estrapolato il costo standard, a dire che il costo della la sanità delle sue Prealpi

di una persona che ha 40-50 anni. Non possiamo fare queste sciocchezze! Per assicurare un servizio uguale a tutti,

tranne il 3). A livello regionale, lei ha accettato la proposta delle piccole Regioni, ed è giusto che sia così, anche se non sono tanto convinto, perché alcune volte ci sono piccole Regioni ricchissime. Comunque, credo

il costo standard e il relativo fabbisogno che viene espresso in funzione del territorio, se dovessimo inserire i parametri indicati dal senatore Astore, dovremmo tenere conto

Presidente, noi voteremo contro questo articolo per le ragioni che sono state illustrate prima. Riteniamo infatti che il sistema di perequazione non garantisca quegli obiettivi a cui ci siamo già riferiti. La conquista nominale del carattere verticale

rispetto alla necessità di verificare e ridefinire, in modo periodico, i canali di finanziamento della perequazione e il meccanismo di calcolo del fabbisogno standard per i livelli essenziali di prestazione.

si parla della «valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni demografiche» e così via, facendo riferimento ai piccoli Comuni e ai territori montani: noi chiediamo di aggiungere anche le isole minori, che sono state aggiunte in altra parte del testo

Presidente,

dal senatore Stradiotto Signor Presidente, con l'emendamento 12.510 proponiamo di inserire al comma 1, dopo la lettera

mattina abbiamo ascoltato tutti quanto ci ha detto il ministro Tremonti, ovvero che il patto di stabilità è cardine rispetto a questo provvedimento sul federalismo fiscale. Con questo emendamento chiediamo che venga espressamente chiesto agli enti locali quello che possono dare e non quello che non possono dare,

vorrei richiamare l'attenzione del Governo su questo emendamento. Cos'è che renderebbe credibile lo sforzo di di implementazione di un sistema federale nel nostro Paese, sforzo che sarà necessariamente lungo, incerto e complesso? Renderebbe credibile questo sforzo la dimostrazione che nelle scelte dell'oggi, non in quelle del domani, si pone grande attenzione sul fatto che i nostri Comuni siano dotati di risorse sufficienti e che l'attribuzione di tali risorse sia legata all'effettiva realtà Se non si fa questo, tutto lo sforzo per rendere credibile il percorso del federalismo rischia di annegare in una contraddizione evidente: domani, forse, il federalismo, oggi il taglio alle autonomie municipali. Questa è una norma che potrebbe essere tranquillamente approvata. Certamente sarebbe, fortemente innovativa, ma darebbe il segno di un vero cambiamento. Non volete approvarla e confermate il rischio che il provvedimento sul federalismo sia più un manifesto di buone intenzioni che la reale trasformazione di cui il Paese avrebbe bisogno.

sul fatto che la compartecipazione all'IRPEF, in una misura che dovrà essere definita, rappresenti uno dei finanziamenti che deve restare in capo agli enti locali. dall'approfondimento fatto in Commissione, si è resa evidente la necessità che vi siano una serie di tributi cui fare riferimento, perché l'ipotesi dell'utilizzo esclusivamente dell'IRPEF determina una sperequazione rispetto al territorio, avendo l'IRPEF una caratteristica di sperequazione. Quindi, il 20 per cento piuttosto che una qualunque altra cifra non dà delle risposte, che possono essere sicuramente condivisibili in certe aree del Paese mentre non determinano un finanziamento adeguato delle risorse in altre. Quindi, il *mix* riteniamo debba essere la formula, tra cui ovviamente anche la compartecipazione all'IRPEF, ma per determinare di partenza una perequazione tale e ricorrere per quanto possibile, il meno possibile, al fondo perequativo. Diversamente, ritorneremmo ad un trasferimento erariale mascherato.

aggiungere la seguente: «*i-bis)* previsione che la legge statale, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali virtuosi» - visto che in un altro articolo di riferimento

previsione che la legge statale, nell'ambito della premialità ai Comuni virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale.».

elementi d'innovazione, dal nostro punto di vista, di miglioramento del testo dell'articolo 12, precisando in maniera più puntuale le basi imponibili cui far riferimento per garantire l'autonomia finanziaria degli enti locali; soprattutto, c'è un'articolazione di elementi che riguardano, ad esempio, la flessibilità dei tributi cui poter fare riferimento. Consideriamo altresì molto importante la compartecipazione

che dovrà fare il Governo per fronteggiare l'andamento critico dell'economia del nostro Paese, liberando risorse che possono essere effettivamente messe a servizio del rilancio con

perché riteniamo che quando s'interviene in attuazione dell'articolo 119, e, in particolar modo, di quella norma costituzionale che prevede

perché è in netto contrasto con il terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione. Com'è noto, questa disposizione costituzionale prevede che il fondo perequativo

per scrivere le norme che dovrebbero garantire il riequilibrio della capacità fiscale per abitante attraverso il fondo perequativo è una forzatura sul piano politico ed istituzionale. Ma l'idea che addirittura il legislatore statale, in sede di delega, possa attribuire per una parte ad un soggetto costituzionalmente non rilevante (cioè le Regioni), ai fini del fondo perequativo, e prevedere che una quota parte del fondo perequativo (cioè quella destinata alle Province e ai Comuni) non solo sia iscritta nel bilancio delle Regioni, ma che queste possano discrezionalmente scostarsi dalle indicazioni statali e stabilire, per la gestione della perequazione, modalità e criteri diversi, quando si tratti di Comuni e Province, mi sembra una cosa che non può stare in piedi.

Il fondo perequativo ha questa funzione. Il legislatore statale non ha neanche la possibilità di variare il criterio, anch'esso costituzionalmente stabilito, che è uno e uno solo, cioè la capacità fiscale per abitante. Allora, cosa si sarebbe dovuto fare? Si sarebbe dovuto riservare alla legge dello Stato e disciplinare in questa sede e in via esclusiva questa materia, poiché la Costituzione dice che questo fondo riguarda le Regioni e gli enti locali, Comuni e Province con minore capacità fiscale. Poiché tutto questo non viene fatto e poiché si fa un'ulteriore forzatura prevedendo che questo fondo sia delegato e appaltato alle Regioni per quanto riguarda la gestione della quota parte destinata a Province e Comuni si fa un doppio errore: il primo sotto il profilo istituzionale e costituzionale e l'altro sotto il profilo politico. Mi scandalizza, signor Presidente, l'assordante silenzio dell'ANCI su questa impostazione. veramente inqualificabile - mi si passi il termine - perché sul piano politico si ripristina il principio del neocentralismo regionale in forza del quale non solo non c'è più un rapporto diretto tra lo Stato e gli enti locali, non solo non si tiene conto dell'autonomia che l'articolo 114 della Costituzione ha dato a Comuni, Province e Città metropolitane, ma in aggiunta a questo si crea una dipendenza ulteriore sotto il profilo economico, al di là delle competenze che la Regione ha nel disciplinare i tributi e le compartecipazioni regionali degli enti locali, e si attribuisce un'ulteriore competenza, una sovranità e un potere di ingerenza delle Regioni oltre quello che la Costituzione prevede. Noi abbiamo provato con alcuni emendamenti a modificare e correggere. Preannunzio, tra l'altro, che ritiriamo gli emendamenti sostanzialmente correttivi di alcune parti

capacità per abitante fiscali standard. Innanzitutto, sul fondo perequativo diviso presso le Regioni tra Province e Comuni

poiché è lo Stato che deve garantire attraverso la perequazione la coesione nazionale - sono due aspetti che si sposano e procedono insieme - ricorrere a questo meccanismo barocco

l'istituzione di un fondo per la perequazione per i Comuni non intestato sul bilancio dello Stato, ma su quello delle Regioni. Quindi, in questa maniera, con tutte le cautele presenti nel testo e che io non voglio disconoscere, in realtà si altera la disposizione centrale della Costituzione. In sostanza, si fa della perequazione non più una funzione fondamentale dello Stato ma una funzione delle Regioni o una funzione compartecipata delle Regioni e dello Stato. Questo mi sembra francamente non proponibile. L'emendamento 13.522 è puramente tecnico. Infatti, se venisse approvato il

L'emendamento 13.525 attira l'attenzione su un tema che era già stato affrontato dal collega Astore nel suo ultimo intervento, cioè la necessità di tener conto in modo adeguato

e modellando il criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. Si tratta di realtà difficili, minori, che non devono essere perse dentro questa grande iniziativa - sperando che riesca - di perequazione.

vogliamo garantire l'eliminazione della differenza fra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ogni ente, perché è evidente che non possiamo penalizzare

Signora Presidente, inizio con una nota di colore relativamente alla cravatta. Sembra che in questa Camera non ci si possa mettere la cravatta verde senza essere automaticamente iscritti al Gruppo della Lega. Si sappia che è la *pochette* nella tasca che fa il leghista, oltre alle cose che si dicono e che si pensano. Il verde mi fa collegare alla bandiera della Libia. Oggi alla Camera è stato approvato il Trattato di amicizia tra l'Italia con grande richiesta da parte di tutti coloro che hanno partecipato al dibattito di una diretta radiotelevisiva sulla emittente pubblica RAI, relativamente se non altro alla parte di dibattito generale. Spero che almeno il Senato riesca a dare prova della possibilità di rendere trasparenti le nostre discussioni relativamente a un accordo che chiede di dare 5 miliardi degli italiani, in una congiuntura economica sfavorevole, a un Governo dittatoriale. trasferirà la sua richiesta alla Conferenza dei Capigruppo e all'Ufficio di Presidenza.

del disegno di legge "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", premesso che